che si pongono molti italiani, sia lavoratori e famiglie, sia (soprattutto) il settore economico. Quindi, non solo gli autotrasportatori, ma anche tutta la piccola e media impresa.

con un retroscena di speculazioni, di interessi privati, di interessi di grandi aziende che ricadono sulle spalle dei piccoli risparmiatori. Ma a parte questo problema, che dovremo discutere la prossima settimana sperando di trattare finalmente la mozione relativa ai mercati finanziari,

il Ministero dello sviluppo economico effettua un regolare monitoraggio dell'andamento dei prezzi dei petroliferi di largo uso attraverso una rilevazione settimanale che tende a verificare, anche attraverso un confronto su base europea, che i prezzi praticati siano adeguati alle oscillazioni del costo del petrolio. Tale costante monitoraggio ha evidenziato un raffreddamento nell'ultimo trimestre 2008 della dinamica dei prezzi, dovuto essenzialmente al calo delle quotazioni del prezzo del petrolio, che ha provocato una diminuzione del costo industriale dei carburanti. La rilevazione sui carburanti del 5 gennaio 2009 ha registrato un ulteriore ribasso, che ha portato la benzina a 1,083 euro a litro e il gasolio a 1,022 euro a litro, con una riduzione rispetto ai valori dello scorso luglio rispettivamente del 40,6 per cento per la benzina e del 48,5 per cento per il gasolio. Circa l'adeguamento dei prezzi dei carburanti all'andamento della quotazione del petrolio si evidenzia che i prezzi dei carburanti seguono nella loro dinamica gli andamenti dei corrispondenti prodotti raffinati (benzina e gasolio) scambiati sui mercati petroliferi internazionali, (rilevati dal Platts) le cui tendenze non sempre coincidono con quelle del greggio e vanno valutate su un periodo di tempo significativo, diverso rispetto alla singola settimana o giorno; i prezzi italiani di benzina e diesel (al netto delle tasse) si sono progressivamente ridotti in linea con gli altri Paesi europei. In dettaglio, da luglio 2008 il prezzo dei carburanti sui listini è sceso allo stesso ritmo, se non in misura maggiore, di quello delle quotazioni internazionali del greggio e dei prodotti raffinati. Sul mercato internazionale di riferimento, la benzina dal 16 luglio al 19 dicembre scorso ha perso 0,329 euro a litro, mentre la componente industriale del prezzo Italia (al netto di accise ed IVA) 0,365 euro al litro e il prezzo Italia alla pompa 0,438 euro a litro. Il diesel invece ha lasciato sul terreno 0,396 euro a litro sul mercato internazionale di riferimento, mentre la componente industriale del prezzo Italia (al netto di accise ed IVA) 0,401 euro al litro e il prezzo Italia alla pompa 0,481 euro a litro. Per quanto riguarda il mercato dei greggi, dopo aver toccato il 3 luglio dello scorso armo il record storico di 144,22 dollari a barile (pari a 0,571 euro a litro) il *brent dated* è crollato a 39,97 dollari a barile (pari a 0,181 euro a litro), il che si traduce in un ribasso di 0,390 euro a litro. Se si raffrontano le riduzioni dei prezzi medi industriali di dicembre con quelli di luglio 2008 nei 15 maggiori Paesi europei, si può notare che nella media UE da luglio a dicembre i prezzi si sono ridotti di 324,5 euro per mille litri sulla benzina e 333 euro sul diesel, mentre in Italia si sono ridotti, rispettivamente, di 324 e di 335,3 euro, quindi perfettamente in linea. dall'inizio del 2009, sulla scia della crisi di Gaza che ha riaperto le tensioni nel mondo arabo e delle attuali problematiche sul fronte gas tra Russia e Ucraina, si è registrato l'avvio di un aumento generalizzato dei prezzi del greggio, che potrebbe dar corso, a breve, a conseguenze sui prezzi carburanti. Sulla differenza della variazione percentuale tra il prezzo del greggio e quello della benzina, va rilevato che la variazione del greggio incide solo sulla componente industriale del prezzo della benzina, non avendo alcun impatto sull'accisa,

del mese di gennaio, rappresenta un indubbio sollievo per i bilanci, soprattutto delle famiglie, pur in un quadro di preoccupazione per il rallentamento dell'economia globale. Anche nei prossimi mesi dovrebbe proseguire la riduzione dei prezzi dei prodotti energetici e delle bollette di luce e gas. Ciò consentirà alle famiglie di spendere meno nel 2009 rispetto ai picchi del 2008. In merito agli interventi del Governo per rendere per i cittadini il prezzo della benzina meno gravoso e più proporzionato al prezzo del greggio, si evidenzia inoltre che dal giugno 2008 è operativo il tavolo permanente di confronto con i petrolieri, istituito per far fronte all'esigenza, attraverso il confronto con gli operatori e le categorie interessate, di trovare soluzioni in grado di incidere sulla struttura del settore e ridurre la distanza del costo industriale dei prodotti petroliferi tra l'Italia e gli altri Paesi europei. L'attività del tavolo, che proseguirà anche nel 2009, è stata orientata nel corso del 2008, tra l'altro, a promuovere il provvedimento di legge per rimuovere alcuni vincoli commerciali all'apertura di nuovi distributori, anche al fine di risolvere il contenzioso comunitario in atto, e a definire una nuova metodologia di analisi dell'andamento dei prezzi. Al riguardo, si evidenzia che con la legge n. 133 del 6 agosto 2008, articolo 83-*bis*, commi 17 e seguenti, si è proceduto anche alla riforma del settore della distribuzione dei carburanti, per rispondere pienamente ai profili contestati dall'Unione europea nella procedura di infrazione 2004/4365, e si è avviato il chiarimento, a livello regionale, dell'immediata ed integrale applicazione della normativa in questione. Alcune Regioni, infatti, hanno già diramato circolari esplicative in tal senso ai Comuni, agli operatori ed a tutti i soggetti interessati. Si evidenzia, infine, che per la rilevazione dei prezzi si è giunti all'adozione di una metodologia di analisi di andamento dei prezzi e del confronto con i 15 Paesi dell'area euro, che tiene conto anche delle promozioni e delle offerte commerciali di benzina e gasolio.

"La Perla S.p.A", azienda storica bolognese, *leader* nel settore dell'intimo, dell'abbigliamento mare e della *lingerie*, è tuttora presente su tre siti produttivi: a Bologna in via Mattei, a Ozzano Emilia e a Granarolo dell'Emilia. Il primo agosto del 2007, la società è stata acquisita dal fondo di *private equity* "JH Partners" che ne ha cambiato la denominazione in "La Perla s.r.l". Il *management* è stato rafforzato con una squadra di dirigenti di livello internazionale, che ha avviato un processo di modernizzazione, con l'obiettivo di favorire una dimensione internazionale del Gruppo. Il nuovo modello organizzativo prevedeva una riduzione degli occupati fino ad un massimo di 365 unità su 735 unità presenti sul territorio bolognese. La vertenza è stata seguita a livello locale. Nel corso dei numerosi incontri svolti, la direzione de "La Perla" ha illustrato la complessiva situazione dell'azienda, presentando alle organizzazioni sindacali un'ampia documentazione contenente le risultanze del *chek-up* economico, finanziario e organizzativo condotto dal nuovo *management* e il piano industriale per il periodo 2009-2010. Nell'ultimo incontro, svolto il 23 dicembre 2008 presso la sede della Provincia di Bologna, presenti i rappresentanti della Provincia di Bologna, della Regione Emilia Romagna, del Comune di Ozzano dell'Emilia, dell'azienda e delle rappresentanze sindacali unitarie, la società ha confermato la volontà di potenziare la presenza dei prodotti "La Perla" sui mercati internazionali attraverso le iniziative dettagliatamente illustrate nel piano industriale, che riguardano ogni area aziendale e sono riconducibili alle strategie commerciali, di prodotto e di processo ritenute necessarie per attuare il riequilibrio economico e il rilancio aziendale. Nel corso del confronto sul piano aziendale, le organizzazioni sindacali hanno valutato positivamente il progetto industriale. Preso atto della necessità di procedere ad una riorganizzazione aziendale finalizzata alla salvaguardia e allo sviluppo dell'azienda, i sindacati hanno chiesto, tuttavia, di porre particolare attenzione ai problemi occupazionali e sociali che potrebbero derivare dall'attuazione degli interventi previsti. Al termine del confronto, le parti hanno concordato di utilizzare lo strumento della Cassa integrazione guadagni straordinaria

con il coinvolgimento in media di 250 lavoratori e che, nel rispetto delle programmazioni previste dal piano industriale, i dipendenti le cui attività siano fungibili professionalmente ed organizzativamente, saranno posti in cassa integrazione a rotazione, per reparto o ufficio, salvaguardando le esigenze tecnico-produttive. Le parti, riconoscendo che la formazione e la riqualificazione professionale sono strumenti atti a favorire la costituzione del nuovo modello di sviluppo e la ricollocazione sia interna che esterna, (con l'obiettivo di affrontare la gestione di eventuali esuberi) hanno altresì convenuto di definire, a breve, i contenuti dei programmi formativi che accompagneranno la riorganizzazione aziendale. Il Ministero dello sviluppo economico vigilerà affinché sia data completa attuazione agli impegni assunti, che dovrebbero consentire all'azienda in questione di riposizionarsi con successo sul mercato, in tempi ragionevolmente brevi.

29 ottobre, nel pieno della crisi di cui il Sottosegretario in questo momento ha dato conto. La mia soddisfazione rispetto alla descrizione degli eventi e allo stato dell'arte della crisi de "La Perla" non può essere

storica, connotata territorialmente, (una famiglia di imprenditori locali che partendo da un'attività artigianale aveva nel tempo sviluppato un'attività a valenza internazionale)

avvenga in termini assolutamente rigorosi e che gli impegni che la proprietà ha preso, che prevedono un investimento di oltre 8 milioni di euro per la riqualificazione aziendale, siano effettivamente mantenuti

fondamentale della Provincia e della Regione, che hanno dichiarato la propria piena disponibilità ad accompagnarlo, sia in termini procedurali sia in termini economici, mettendo a disposizione risorse e strumenti per i piani di formazione e di riqualificazione delle addette, delle addette, che dovranno essere ricollocate, sia nel nuovo impianto produttivo sia, eventualmente, come veniva ricordato, all'esterno dell'azienda. Chiedo che il processo venga attentamente monitorato e seguito, perché due anni di cassa integrazione straordinaria sono un'occasione irripetibile per recuperare una realtà che per il territorio di Bologna e dell'Emilia-Romagna è fondamentale, soprattutto in ordine all'occupazione femminile. Concludo richiamando un altro aspetto che mi pare fondamentale. Il Partito Democratico in questi ultimi mesi ha più volte indicato la necessità di intervenire con misure non ordinarie di fronte a questo stato di crisi. L'utilizzo, come in questo caso, della cassa integrazione straordinaria come strumento per risolvere

più ricche a livello nazionale e l'utilizzo degli strumenti straordinari è aumentato in un anno del 573 per cento. Invito quindi il Governo a riflettere approfonditamente, anche in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 1167, in discussione al Senato, su una piena e totale revisione degli strumenti di accompagnamento delle crisi industriali e di supporto all'occupazione.

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni in esame, trattando le stesse del medesimo argomento. Il protocollo d'intesa tra il Governo e la Regione Basilicata, sottoscritto il 7 ottobre 1998, riguarda un piano di interventi diretti ad accelerare lo sviluppo socio-economico delle aree della Regione Basilicata interessate all'estrazione di idrocarburi. In particolare, tale documento prevede la realizzazione di una serie di interventi infrastrutturali, nonché impegni per la realizzazione del programma di completamento della metanizzazione e di sviluppo dei giacimenti petroliferi della Regione Basilicata. Al fine di controllare l'attuazione degli impegni assunti il citato protocollo prevede, inoltre, la costituzione di un comitato paritetico, composto da sei membri in rappresentanza delle amministrazioni centrali e della Regione Basilicata e presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per l'individuazione delle misure di rilancio dei programmi di industrializzazione della Val Basento è previsto un apposito tavolo di lavoro costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto riguarda lo stato di attuazione degli impegni assunti con il predetto protocollo, si segnala che il programma di metanizzazione relativo ai progetti, oggetto di intervento ai sensi della legge n. 266 del 1997, è stato regolarmente attuato ed è in corso di ultimazione.

Il progetto di sviluppo dei giacimenti della Val d'Agri è stato condotto a termine, seppur con ritardo, ed alcune incompletezze riscontrate nella realizzazione delle infrastrutture non hanno finora consentito la piena valorizzazione delle risorse presenti nel sottosuolo. Attualmente, il Centro olio della Val d'Agri risulta regolarmente in funzione e produce circa 3,6 milioni di tonnellate di petrolio e 1,2 miliardi di metri cubi di gas metano all'anno. Per quanto riguarda, invece, lo stato di attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione Basilicata ed ENI, occorre evidenziare che si tratta di un documento finalizzato non solo allo sviluppo delle attività petrolifere, ma anche al rilancio dello sviluppo economico e sociale della Regione stessa, traendo spunto e risorse finanziarie anche dalla programmata coltivazione delle risorse petrolifere rinvenute nella Val d'Agri. Tale documento prevede, infatti, opere di compensazione territoriale, monitoraggio ambientale, formazione professionale e sviluppo in loco dell'indotto, sviluppate con 11 accordi attuativi, siglati dai medesimi soggetti che riguardano: la compensazione ambientale; il sistema di monitoraggio ambientale; 1'estensione della rete metano; l'Osservatorio ambientale; le borse di studio; la Fondazione Enrico Mattei; lo sviluppo sostenibile; la gestione del monitoraggio ambientale; la Società regionale per l'energia; l'Agenzia per lo sviluppo; l'anticipazione delle *royalties* future. L'insieme delle misure previste dal protocollo comportava una spesa pari a 180 milioni di euro. Ad oggi, risulta che l'ENI abbia erogato circa 85 milioni di euro alla Regione, circa 1,5 milioni di euro alla Fondazione Enrico Mattei e circa 0,5 milioni di euro all'Osservatorio ambientale. Si può dire, pertanto, che gli interventi previsti sono stati attuati nella misura del 48 per Da informazioni acquisite presso l'ENI, risulta che le attività relative alla compensazione ambientale, al sistema di monitoraggio ambientale, all'estensione della rete metano, all'Osservatorio ambientale, alle borse di studio e alla Fondazione Enrico Mattei sono in corso di attuazione, mentre quelle relative allo sviluppo sostenibile ed alla gestione del monitoraggio ambientale non possono ancora essere attuate, in quanto ricorrono delle condizioni sospensive (si è in attesa infatti di alcune autorizzazioni). Le attività relative alla Società regionale per l'energia, all'Agenzia per lo sviluppo e all'anticipazione delle *royalties* future non sono ancora state attuate, in quanto risulterebbero ancora in corso di definizione aspetti di dettaglio. Per quanto riguarda la richiesta di una riduzione delle accise sui carburanti a favore della popolazione della Basilicata, si precisa quanto segue. La disciplina delle accise, nel prevedere il sorgere dell'obbligazione tributaria al momento della fabbricazione (o dell'importazione) dei prodotti sottoposti ad accisa, ne procrastina l'esigibilità al momento dell'immissione al consumo dei medesimi e consente, ai sensi della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, l'applicazione di un'aliquota ridotta o di un'esenzione solo nel caso in cui i prodotti tassati vengano impiegati in alcune specifiche attività. Ciò precisato, si fa presente che il Governo, al fine di favorire i residenti nelle Regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ha presentato proposta di emendamento all'articolo 27 dell'Atto Senato n. 1195, attualmente all'esame della 10a Commissione finalizzato alla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine. Tale emendamento prevede che per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi, ottenute in terraferma a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sia elevata dal 7 per Le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota sono destinate esclusivamente al Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per i residenti nelle Regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Per quanta riguarda, in particolare, il quesito posto dal senatore Latronico in merito alle «istanze di concessione di coltivazione di idrocarburi e allo stato delle procedure relative al conferimento dei titoli minerari», si fa presente che attualmente non risulta essere stata presentata nessuna nuova istanza di concessione di coltivazione di idrocarburi ricadente in tutto o in parte nel territorio della Regione Basilicata. Risultano, invece, in fase istruttoria, d'intesa con la Regione medesima, 28 istanze relative a permessi di ricerca. A tal proposito si evidenzia che lo stato delle procedure è differente per ogni singolo caso

alla mancanza di espressione di intesa da parte della Regione interessata. In Basilicata insistono, inoltre, 23 permessi di ricerca e 21 concessioni di coltivazione già conferiti. Infine, si segnala che soltanto per alcuni dei suddetti titoli minerari sono regolarmente in svolgimento le attività approvate d'intesa con la Regione, a causa di difficoltà legate all'acquisizione delle autorizzazioni in sede locale.

Considerato che la Regione Basilicata rappresenta il più grande produttore di petrolio *onshore* in Europa - mi pare che siamo l'ottava area petrolifera del mondo per estrazione petrolifera - e che

rispetto alle esigenze delle nostre popolazioni che richiedono un utilizzo congruo delle risorse naturali che fanno parte del sottosuolo della nostra Regione. La risposta del Governo con l'emendamento citato dal sottosegretario Romani è puntuale perché attiene ad una richiesta ben precisa fatta

Quell'emendamento rientra in maniera precisa in questa direzione e ringrazio, ancora una volta, il Governo per l'attenzione e la sensibilità dimostrata verso questo tema. Vorrei anche sottolineare, come si evince da quello che

anche nella risposta del Sottosegretario, che la Basilicata rappresenta un potenziale produttivo per quanto riguarda l'estrazione mineraria straordinariamente importante per tutto il Paese.

che non può più attendere. I numeri sono eloquenti: ci sono altre 28 istanze di permessi di ricerca, che si aggiungono ai 23 permessi già concessi e alle 21 concessioni già conseguite. L'intero territorio della Basilicata Basilicata ha un potenziale straordinario per i fabbisogni energetici dell'intera Nazione, ma questa comunità regionale si attende le ricadute che dieci anni fa il Governo regionale, il Governo nazionale e le concessionarie hanno sottoscritto. A fronte di una disponibilità territoriale e ambientale straordinaria, i lucani si attendevano e si attendono ricadute dirette sul proprio sviluppo, quindi parliamo di un risarcimento per consentire a quelle popolazioni di mettere in moto un processo di autosviluppo. Pertanto non possiamo che apprezzare, signor Sottosegretario, suo tramite, l'opera del Governo perché, qualora l'atto Senato n. 1195, cui si riferisce l'emendamento del Governo, del Governo, incrementasse le *royalties,* come lei ha annunciato, del 3 per cento per istituire un fondo per l'abbattimento del prezzo delle benzine, daremmo una prima risposta a questa domanda di risarcimento. Ovviamente, poi, impegniamo il Governo affinché tutte le parti nobili dell'accordo sottoscritto con l'ENI, quelle che riguardano appunto lo sviluppo delle attività produttive della Regione Basilicata, siano onorate.

economico*. È da segnalare, innanzitutto, che il «catasto nazionale delle frequenze» è ormai una realtà operativa al servizio degli operatori di comunicazione. Per la sua realizzazione, il censimento degli impianti radiotelevisivi è stato preventivamente effettuato su tutto il territorio, compresa la Regione Campania. Una nuova modalità di gestione del *database*, attraverso l'utilizzo della rete Internet ha, inoltre, reso più agevole l'implementazione del catasto da parte degli operatori e la consultazione dei dati in esso contenuti, compresi, ovviamente, quelli relativi alle emittenti che operano in Campania. Il sistema consente oggi a ciascun operatore di disporre *on line* dei dati tecnici dei propri impianti radioelettrici e di effettuarne i relativi aggiornamenti, attraverso tecniche di tracciamento degli accessi al *database* che consentono anche di ricostruire la storia di ciascun impianto. Sotto il profilo dei controlli radioelettrici, poi, la costituzione del «catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive» ha rappresentato, per gli organi preposti alle verifiche, un utile strumento per mettere in atto un'azione più incisiva sul territorio e per far emergere l'abusivismo degli impianti radioelettrici, fenomeno più o meno diffuso in molte Regioni italiane. In concreto, negli anni passati, è stata avviata dall'ex Ministero delle comunicazioni (oggi dello sviluppo economico), in collaborazione con gli Ispettorati territoriali competenti, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Sezione di polizia postale e delle comunicazioni, una campagna di controlli e di riscontri tecnico-amministrativi su tutto il territorio nazionale nei siti di particolare interesse radioelettrico. Lo scopo di tali controlli era mosso dalla necessità di verificare la corrispondenza delle dichiarazioni effettuate dai vari operatori, relativamente agli impianti da loro dichiarati in sede di primo censimento. Nel corso del 2008, tale attività di verifica è stata svolta anche nella Regione Campania, ad opera dell'Ispettorato territoriale in collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni. in particolare, in data 29 aprile 2008 è stata effettuata una serie di sopralluoghi tecnici congiunti anche agli impianti radioelettrici installati nei pressi del Monte Faito, che irradiano il segnale nel bacino della Regione Campania e, soprattutto, nella città di Napoli. Si può quindi affermare che anche in Campania il sistema delle radiofrequenze non è sfuggito al controllo e che, anzi, attraverso una capillare azione sul territorio, gli accertamenti sono stati intensificati al di là delle normali verifiche di *routine*. Dai dati comunicati dagli uffici preposti al controllo, si segnalano: 659 sopralluoghi presso punti territoriali di particolare interesse radioelettrico, destinati all'esame di parametri tecnici del segnale radiotelevisivo emesso dagli impianti degli operatori; 97 interventi volti a trovare i soggetti responsabili di turbativa alle comunicazioni; 23 richieste di applicazione dell'articolo 195 dell'ex codice postale inerente l'installazione o l'esercizio abusivo degli impianti radioelettrici, per la cui violazione è previsto il sequestro penale degli stessi apparati; 31.625 controlli tecnici effettuati dalle postazioni fisse di monitoraggio elettronico e automatico, dislocati in ciascuna sede provinciale della Regione Campania. Per tenere sotto controllo tale delicata situazione il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, attraverso il competente Ispettorato territoriale, in collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni, si farà cura di intensificare comunque le verifiche degli impianti radiotelevisivi nella Regione, anche ai fini della pianificazione delle frequenze in digitale, in previsione dello *switch off* nell'area previsto alla fine del 2009. Per quanto riguarda il secondo quesito posto dagli interroganti, in merito ai provvedimenti diretti a porre termine al regime di *prorogatio* del CORERAT Campania, si informa che con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 235 del 27 novembre 2008, è stato istituito il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM). Lo stesso decreto ha provveduto alla nomina del Presidente e degli otto componenti del Comitato. L'organismo si è insediato ed è già operativo. Per quanto concerne, infine, la propaganda culturale di prossimità con il sistema camorristico, la questura di Napoli ha comunicato che allo stato, da indagini effettuate, non risultano elementi in merito. In ogni caso, anche alla luce dell'interrogazione cui si fornisce la presente risposta, potranno essere disposte ulteriori verifiche.

come proprietario di emittenze e in rapporti dubbi con il sistema camorristico, è stato arrestato nell'ottobre 2008 nell'operazione "Onde rotte", il cui titolo è già abbastanza espressivo, coordinato dal sostituto procuratore Aldo De Chiara, che ha portato all'esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari per Giuseppe Giordano, la moglie Domenica Sarnataro, legale del rappresentante della "Italia mia Group Spa", cioè la emittente, detentrice dell'emittente "Italia mia", il figlio Ciro Giordano ed il nipote Ciro Giordano. Si potrebbe attestare una dimensione un po' vernacolare della comunità familiare, ma la cosa risulta abbastanza preoccupante proprio perché questo Ciro Giordano è ormai, in modo evidente, in connessione con il sistema camorristico. La questione del CO.RE.COM è a sua volta da monitorare con attenzione perché il CO.RE.COM. campano avrebbe elargito contributi, ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 448 del 1998, per emittenti locali pari a 10 milioni di euro l'anno, a quanto pare senza canoni stringenti sulla qualità editoriale. Per concludere, è desiderabile che vi siano sistemi di indagine aggiornati su tutti questi fenomeni di diffusione delle reti, reti, ma ci vorrebbe anche un'attenzione specifica rivolta a cercare di capire quanto il sistema della criminalità organizzata possa essere in

che nella Regione Campania l'emittenza fiancheggiatrice degli spunti camorristici arriva addirittura a rappresentare in modo

poiché si tratta di un sistema di diffusione televisiva, senza per questo accedere all'idea che si debba praticare la censura, perlomeno, un'attenzione vigile su fenomeni di questo tipo potrebbe essere forse condotta e di ciò non trovo traccia nella risposta del Sottosegretario.

Signora Presidente, la questione riguarda la richiesta di sospensione temporanea delle procedure di vendita del complesso denominato Villaggio Santa Barbara, in attesa di ricevere chiarimenti da parte dell'Agenzia del demanio in merito alle condizioni di vendita, e, in specie, sulla corrispondenza del prezzo di vendita proposto agli inquilini con il reale valore degli alloggi. Al riguardo, si fa presente che l'Agenzia del demanio ha fornito chiarimenti in merito alle osservazioni formulate dai senatori interroganti, dando risposta con nota (protocollo n.

non può che rendersi noto che in quell'anno le operazioni di vendita non ebbero corso in quanto il compendio in parola era ancora in uso governativo al Ministero dell'interno e come tale appartenente al patrimonio indisponibile. Essendosi perfezionate le procedure di dismissione dall'uso governativo soltanto nel corso dell'anno 2003, ed avendo dovuto l'Agenzia procedere, ai fini della futura vendita degli alloggi in parola, ad una complessa e prolungata attività di regolarizzazione

Pertanto, questa Agenzia ha proceduto alla determinazione del valore di mercato di ciascuna unità immobiliare attraverso il metodo sintetico-comparativo. Tale metodo prevede la comparazione con immobili, appartenenti alla tipologia residenziale, assimilabili a quello oggetto di valutazione per caratteristiche intrinseche (consistenza, stato manutentivo, eccetera) ed estrinseche (ubicazione, collegamenti, eccetera). Da tale procedimento è stato ricavato un valore unitario riferito al metro quadro di superficie lorda compreso all'interno dell'intervallo indicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio per il secondo semestre 2006. I valori unitari sono stati poi moltiplicati per la superficie lorda dei singoli alloggi, determinando il valore di mercato di ciascuno degli appartamenti. II prezzo di acquisto delle unità immobiliari indicato nelle proposte di vendita è stato determinato detraendo dal valore di mercato, individuato per ogni unità, una percentuale pari al 30 per cento, in conformità con quanto previsto dalla citata legge n. 662 del 1996. Si precisa, inoltre, che il comma 256 dell'articolo 1

aggiungendo un periodo al comma 219 della legge n. 296 del 2006, che conferma l'attribuzione all'Agenzia del demanio, a seguito della soppressione, ai sensi del decreto legislativo n. 300

Giova far presente che la correttezza dell'operato dell'Agenzia e l'equità del prezzo determinato per la cessione degli alloggi in parola sono confermate dall'avvenuta vendita di 14 unità immobiliari occupate con regolare pagamento in favore degli inquilini e di 2 alloggi liberi, alienati a seguito di procedura ad evidenza pubblica. In ordine al distacco delle utenze degli alloggi dall'adiacente caserma della Scuola di formazione di base dei Vigili del fuoco si precisa che Roma Capitale sta provvedendo, a spese dell'Agenzia, al rifacimento di tutto l'impianto elettrico. Restando a disposizione per ogni ulteriore eventuale richiesta di chiarimenti, si porgono cordiali saluti". Questa era la comunicazione dell'Agenzia del demanio. Per completezza, occorre rappresentare che l'Agenzia del demanio di recente ha comunicato di aver proceduto, nel corso del 2008, alla vendita di talune delle unità immobiliari del compendio di cui trattasi. su un totale di 117 beni si è conclusa la vendita di 26 immobili, di cui 4 alienati tramite asta pubblica ed altre vendite sono previste nel corso del 2009. La stessa Agenzia ha, infine, precisato che per quanto attiene agli immobili non optati non è prevista l'alienazione e, pertanto, i rapporti con gli inquilini continueranno ad essere regolati dal contratto di locazione in essere.

questione è di rilevanza ridotta: siamo in presenza di 136 alloggi di un complesso dei Vigili del fuoco nella zona Sud di Roma, Capannelle. il 1948 e il 1951 in economia - come suol dirsi -dagli stessi Vigili del fuoco, con materiali di risulta dei loro interventi, e quindi hanno una valenza ed un valore di mercato ultrapopolare. Credo che

Le attuali disposizioni normative attribuiscono al prefetto territorialmente competente il potere di sostituire, nei casi espressamente disciplinati, l'amministrazione inadempiente mediante un commissario che provvede d'ufficio agli adempimenti di legge. Peraltro, qualora vi sia fondato motivo di ritenere gli atti illegittimi, l'ordinamento contempla la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Per quanto riguarda il caso specifico del Comune di Ferrandina, dagli elementi forniti dalla prefettura di Matera, risulta che il 23 maggio 2008 il Presidente del Consiglio comunale informava la stessa prefettura di aver convocato il Consiglio, il 31 maggio 2008 in prima convocazione II 4 giugno, un consigliere comunale segnalava alla predetta prefettura la mancata approvazione del bilancio. Conseguentemente, l'Ufficio territoriale del Governo invitava, con provvedimento del 6 giugno 2008, il Consiglio di quel Comune ad adottare, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, il documento contabile stesso, pena la nomina di un Commissario *ad acta*, in caso di inerzia, e l'avvio delle procedure di scioglimento dell'organo. Dette procedure non sono state poi adottate per l'avvenuta approvazione dei documenti contabili il 9 giugno 2008. L'articolo 106 dello Statuto del Comune di Ferrandina disciplina la mancata approvazione dei bilanci nei termini di legge, prevedendo una specifica procedura per la nomina del commissario. Il Sindaco, infatti, ricevuta la comunicazione da parte del segretario comunale della decorrenza dei termini per l'approvazione del bilancio, è tenuto a convocare, entro 48 ore lavorative, la Giunta comunale per nominare il commissario. In caso di inadempimento del sindaco o della giunta il segretario comunale deve informare il prefetto affinché disponga il commissariamento. Al riguardo, la prefettura ha fatto presente che il segretario comunale, contravvenendo alle disposizioni dell'articolo 106 dello Statuto, non avrebbe comunicato al Sindaco e al Presidente del Consiglio la decorrenza dei termini per l'adozione del bilancio al fine di dare successivo corso alla nomina, da parte della giunta, di un commissario per la predisposizione dello schema e l'approvazione del bilancio. Quest'ultimo, secondo l'esposto presentato dalla minoranza consiliare in prefettura il 23 settembre 2008, sarebbe stato competente alla convocazione del consiglio per l'approvazione del bilancio per cui l'avvenuta convocazione dell'assemblea da parte del Presidente del Consiglio era da considerarsi illegittima. Peraltro, non essendo stato proposto alcun ricorso nei termini di legge, l'atto si è consolidato. Ricordo, infine, che la giurisprudenza amministrativa stabilisce che la legge ricollega all'inosservanza del termine di approvazione dello schema di bilancio la semplice apertura di un procedimento sollecitatorio e non la possibilità di avviare una procedura di scioglimento dell'organo. Infatti, come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, con sentenza del 19 febbraio 2007, il presupposto per disporre lo scioglimento dell'ente non è costituito dalla mera inosservanza del termine, ma discende dalla constatata inadempienza ad un'intimazione puntuale e ultimativa dell'organo competente, che attesta l'impossibilità o la volontà del Consiglio di non approvare il bilancio. Il ricorso alla misura dissolutoria, per non invadere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta dell'ente locale, deve costituire l'*extrema ratio* cui far ricorso, dopo aver esperito, con tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento giuridico, ogni utile iniziativa per riportare l'organo al normale funzionamento.

che è stato denunciato dalla minoranza del Consiglio comunale di Ferrandina, ma che segnala una modalità operativa che non sempre soddisfa sia esigenze di legge, sia esigenze di buon funzionamento. Nel caso di specie, come è stato rilevato, in contrasto con la normativa statutaria, il Presidente del Consiglio comunale di Ferrandina ha disposto la convocazione del Consiglio medesimo per l'approvazione del bilancio oltre i termini previsti dalla legge e si ritiene, da parte della minoranza, che questa sia una illegittimità che travolge e invalida la stessa seduta del Consiglio comunale, ritenendo che alla stessa convocazione dovesse provvedere un commissario, come prevede lo Statuto. È una violazione che non è stata impugnata con

il 6 marzo 2008, il segretario comunale di Tursi comunicava alla prefettura di Matera le dimissioni di nove consiglieri comunali su sedici assegnati, assicurando, il giorno successivo, che le firme dei dimissionari erano state tutte apposte in sua presenza. Il Sindaco ed il presidente del Consiglio comunale, con nota del 13 marzo 2008, eccepivano che le citate dimissioni erano illegittime, per la violazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2004, in quanto le stesse non erano state presentate personalmente al protocollo dell'ente comunale e quindi necessitavano di autentica della firma. Sempre in data 13 marzo, il segretario comunale, su richiesta della prefettura di Matera, comunicava "che i nove consiglieri dimissionari si erano personalmente presentati, la sera del 5 marzo, nella propria abitazione, per sottoscrivere le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, con espressa delega al consigliere Annibale Santagata,

La prefettura, in base agli atti acquisiti, il successivo 14 marzo, rappresentava che le dimissioni difettavano sia del requisito della presentazione personale che di valido atto di delega, rilasciato a terza persona e debitamente autenticato. In data 14 marzo, gli stessi nove consiglieri comunali presentavano, al protocollo dell'ente, nuove dimissioni. Intanto il Consiglio comunale di Tursi, ritenendo valide le sole dimissioni del consigliere Santaganta perché presentate personalmente al protocollo dell'ente il 6 marzo 2008 - provvedeva, con delibera del 15 marzo 2008, alla surroga del medesimo. Il 17 marzo 2008, il prefetto di Matera disponeva la sospensione del Consiglio comunale di Tursi, in attesa dell'adozione del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica e nominava un commissario per la provvisoria gestione dell'ente. Avverso il decreto prefettizio, il Sindaco di Tursi ha proposto ricorso al TAR Basilicata il quale, dapprima con decreto n. 133/08 del 18 aprile 2008 e successivamente con ordinanza n. 162 dell'8 maggio, ha accolto la domanda sospensiva. Nel merito, il TAR con sentenza del 20 novembre 2008 ha annullato il decreto del prefetto di Matera del 17 marzo 2008. Parallelamente, avverso la delibera di surroga del consigliere Santagata, è stato proposto ricorso al TAR Basilicata il quale, con ordinanza n. 163 dell'8 maggio 2008, ha respinto la domanda incidentale di sospensione. Successivamente, invece, il Consiglio di Stato, al quale era stato proposto appello contro la citata ordinanza del TAR, con ordinanza dell'8 luglio 2008, ha accolto l'istanza di sospensiva. Il TAR ha quindi emesso, in data 20 novembre 2008, la sentenza dì primo grado n. 952/08, respingendo il ricorso. Allo stato, pertanto, la surroga del consigliere Santagata deve considerarsi legittima. Dopo la sospensiva disposta dal TAR Basilicata del provvedimento prefettizio, l'amministrazione comunale reinsediata procedeva, il 23 aprile 2008, alla surroga degli ulteriori otto consiglieri dimissionari. Il TAR, dopo aver rinviato il ricorso avverso la surroga del consigliere Santagata e quello contro la convocazione del consiglio per la surroga degli otto consiglieri, con la sentenza del 20 novembre 2008, li ha respinti, ed ha respinto, altresì, il ricorso incidentale, volto a conseguire comunque lo scioglimento del consiglio comunale, in forza delle successive dimissioni presentate il 14 marzo 2008. Ciò premesso, questa Amministrazione non può adottare alcun provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico degli enti locali, anche perché non si è mai raggiunto il *quorum* utile per lo scioglimento del consiglio comunale, che il citato articolo prevede in metà più uno dei membri dell'organo consiliare.

Si è in presenza di una dimissione della maggioranza dei consiglieri comunali, 9 su 16. Tra l'altro, si sono dimessi non una volta, ma più volte, finalizzando tali dimissioni non alla loro surroga, come in realtà è accaduto, ma allo scioglimento del Consiglio comunale.

non soltanto non hanno raggiunto lo scopo per cui si sono dimessi, cioè lo scioglimento, ma sono stati finanche surrogati. Ora, di fronte a questa plateale infrazione, non solo della legge ma anche della volontà popolare, credo che il Ministero dell'interno abbia il dovere di fare un approfondimento e di assumere gli atti conseguenti.

Signora Presidente, onorevoli senatori, ricordo preliminarmente che la sicurezza e la tutela dei cittadini rappresentano una priorità assoluta del Governo, da perseguire con tutti i mezzi a disposizione. Il controllo del territorio costituisce un efficace sistema di prevenzione dell'illegalità, notevolmente incrementato negli ultimi mesi attraverso l'emanazione di specifiche disposizioni di legge, che hanno consentito la presenza delle Forze armate nelle aree considerate a maggior rischio. Il concorso dei militari ha comportato un migliore impiego delle forze dell'ordine, con risultati considerevoli. Nel periodo compreso tra il 4 agosto e il 28 dicembre 2008, nelle diverse città dove sono stati impiegati i militari, tra cui Napoli, sono state identificate 134.373 persone e ne sono state denunciate in stato di arresto 417; sono state effettuate 1.218 perquisizioni, 44.354 controlli e 1.711 sequestri di veicoli. Si è proceduto anche al sequestro di stupefacenti, armi e materiale contraffatto, al ritiro di patenti e al controllo di esercizi commerciali. Anche l'estensione del potere del sindaco del potere del sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano, oltre all'incolumità pubblica, anche la sicurezza urbana ha inteso consentire un più efficace controllo del territorio. La maggiore partecipazione del sindaco alla tutela della sicurezza si concretizza anche in una più incisiva cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno. Analoga collaborazione tra le Polizie è garantita sia per quanto attiene i piani coordinati di controllo del territorio, sia per quanto riguarda l'accesso al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, in ordine ai veicoli rubati o rinvenuti. Fino al 31 dicembre 2008 sono state emanate 335 ordinanze da parte dei sindaci, secondo le nuove disposizioni normative. Sotto il profilo tecnico, l'implementazione e la valorizzazione dei sistemi di videosorveglianza contribuiscono a garantire un efficace controllo del territorio, rientrando a pieno titolo tra gli obiettivi prioritari dell'azione di Governo. In collaborazione con le amministrazioni regionali e locali, presso la questura di Napoli, è stato costituito un sistema di videosorveglianza di alcune aree territoriali del capoluogo, condiviso con il comando provinciale dell'Arma dei carabinieri. Il sistema si compone di circa 110 telecamere orientabili e fisse che assicurano, attraverso collegamenti dedicati

Il sistema denominato "Vomero Lungomare" è funzionante dallo scorso mese di settembre, presso le sale operative della questura e del comando provinciale dei Carabinieri di Napoli. Esso consente, oltre alla visualizzazione e alla registrazione delle immagini, anche l'attivazione di allarmi presso le centrali operative delle forze dell'ordine al passaggio dei veicoli segnalati. Il sistema "Vomero Alto", con identiche funzionalità, è stato completato e sono in corso gli adempimenti amministrativi necessari a consentirne l'operatività. [DE Signora Presidente, signor Sottosegretario, sono perfettamente sicura che la situazione dal punto di vista dell'ordine pubblico a Napoli sia notevolmente migliorata:

il lungomare. Napoli è una grande città in cui imperversano bande di ogni genere, di delinquenza giovanile, di scippatori, di rapinatori, che non agiscono sul lungomare o solamente al Vomero. Peraltro, non mi risulta che il sistema

nel 2007 il nuovo sistema integrato di videosorveglianza territoriale intelligente. Non mi pare che in questi anni, da 2003 al 2009, si sia

già in data 4 luglio 2008 il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali è intervenuto a seguito di notizie di stampa concernenti alcune frodi nel settore lattiero-caseario e sulle quali la Guardia di finanza, nel corso degli anni 2006-2007, ha condotto una indagine specifica su disposizione dell'autorità Nello stesso mese di luglio è stato disposto un intervento del comando carabinieri per la tutela della salute (NAS) nei confronti di tutte le ditte che hanno intrattenuto rapporti commerciali con quelle oggetto indagine da parte della procura ed è stato richiesto che analoghe verifiche venissero effettuate presso gli stabilimenti presenti in altri Paesi comunitari. Preciso che, relativamente al settore lattiero-caseario, i NAS nel 2008 hanno effettuato 2.477 ispezioni, rilevando 374 infrazioni di carattere penale e 1.952 di natura amministrativa, che hanno portato alla chiusura di 57 strutture per ragioni Sono state inoltre disposte ispezioni congiunte tra il Ministero e le Regioni presso gli stabilimenti del settore, che prevedono, tra l'altro, la verifica delle procedure dei servizi responsabili del controllo ufficiale. A seguito delle notizie di stampa del 14 ottobre 2008, concernenti la ditta Galbani, il Ministero nella stessa data ha disposto un'ispezione, effettuata congiuntamente dai NAS e dai servizi veterinari della Regione Umbria, dalla quale è emerso che le condizioni igienico-sanitarie della struttura rientrano nella norma; l'ispezione non ha rilevato irregolarità concernenti la contraffazione delle date di scadenza dei prodotti. Sono tuttora in corso accertamenti dei NAS in altri stabilimenti collegati; peraltro non sono stati finora rilevati elementi di rischio per la salute pubblica che possano costituire motivo In Umbria, la ditta Galbani non ha stabilimenti di produzione, ma solo due piattaforme di distribuzione, (Ponte San Giovanni) e a Terni; presso tali centri sono raccolti e distribuiti i prodotti provenienti quotidianamente da un deposito di Roma, che dal 1° gennaio effettua per conto della Galbani la distribuzione di prodotti anche di altre aziende. hanno precisato che presso tale azienda di Roma non viene effettuato stoccaggio prolungato, che dall'accertamento è risultato che nessun prodotto presentava date di scadenza superate e che le etichettature non mostravano alcun segno di alterazione o manomissione.

nell'interno dello stabilimento in Provincia di Perugia. È quindi attenta la risposta del Governo, ma intenderei conoscere quali sono le attività poste in essere dalla Regione competente sul piano territoriale e dal Ministero competente per ciò che è avvenuto negli anni 2000-2005. Vi è infatti una dichiarazione precisa:

potessero andare in giro. Non devo ricordare a lei che uno degli *slogan* degli anni passati fu proprio: «Galbani vuol dire fiducia»; se la fiducia è quella di ritargare i formaggi per poi portarli in giro... Voglio ricordare anche che numerosi

perché il pericolo riguarda la salute. La fiducia senza dubbio Galbani l'ha persa ritargando i suoi formaggi e i suoi avanzi nel lontano 2005 nella Provincia di Perugia.

sociali*. La questione relativa alla imputabilità degli oneri per le visite fiscali nel pubblico impiego - e, segnatamente, nel settore della scuola - risulta ancora in via di approfondimento, Infatti, pur essendo corretto quanto rilevato dagli interroganti in merito alla sentenza con la quale la Corte di cassazione ha negato la sussistenza del principio della gratuità delle visite fiscali (ci si riferisce alla 13992 del 28 maggio 2008), occorre tuttavia tener conto che la Suprema corte non ha indicato su quale ente debba ricadere il relativo onere finanziario. Al riguardo, si segnala che i competenti Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro, salute e politiche sociali si erano in passato già espressi sulla questione, riconoscendo che gli oneri delle visite fiscali effettuate nei confronti dei pubblici dipendenti sono a carico del Servizio sanitario nazionale. In particolare, il Ministero della salute ha comunicato agli uffici del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in occasione di una precedente interrogazione di analogo oggetto (interrogazione a risposta immediata dell'onorevole Melchiorre 3-00287), di aver sempre sostenuto l'insussistenza di pretese creditorie da parte delle ASL per l'esecuzione delle visite fiscali ai dipendenti pubblici assenti dal servizio per motivi di salute. Ciò sulla scorta di quanto affermato dal Consiglio di Stato, sia in sede consultiva (pareri dell'adunanza generale dell'11 ottobre 1984, sezione seconda del 24 novembre 1993, commissione speciale del 26 ottobre 1994, n. 17, commissione speciale 22 giugno 1995, n. 52), sia in sede giurisdizionale (decreto n. 1909 del 23 dicembre 1998, con il quale è stato respinto l'appello della Regione Umbria avverso una decisione del TAR dell'Umbria). Tale orientamento è stato pienamente condiviso dal Ministero dell'economia e delle finanze per il quale, infatti, l'onere delle visite risulta essere stato posto a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale, con la contestuale soppressione degli specifici capitoli di spesa e degli stati di previsione delle singole amministrazioni e il trasferimento delle somme all'uopo stanziate nel Fondo sanitario nazionale. nel Fondo sanitario nazionale. nell'allegato 1, riporta esplicitamente le «Certificazioni sanitarie ai dipendenti pubblici assenti dal servizio per motivi di salute» tra le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza e già, pertanto, finanziate con le risorse complessive messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale. Il citato provvedimento è stato adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ma ciò non ha impedito che numerose amministrazioni regionali adottassero delibere che ponevano a carico delle amministrazioni richiedenti le spese delle visite fiscali. La sentenza del TAR Lazio n. 4353 del 2004 e, successivamente, la sentenza del TAR Toscana n. 2822 del 2006 hanno poi riaperto i termini della questione, ridando spazio alle richieste di pagamento delle visite da parte delle ASL. Sebbene il Governo e le Regioni abbiano convenuto che fossero necessari ulteriori approfondimenti, il tavolo di monitoraggio e verifica dei livelli di assistenza, attivato presso la segreteria della Conferenza Stato-Regioni, non ha condotto a conclusioni condivise dai diversi soggetti istituzionali partecipanti (Dipartimento della funzione pubblica, Ministero dell'economia, Ministero della difesa, Ministero della salute, Regioni); pertanto, in tale sede si è convenuto di sottoporre le possibili soluzioni evidenziate alla valutazione della Conferenza Stato-Regioni la quale, tuttavia, si è limitata a prendere atto del documento. Sul punto si aggiunge che, come comunicato dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, anche la commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - istituita presso il medesimo Ministero - ha approfondito la problematica di cui trattasi ha approvato, nel 2006, un parere in merito alla attuale disciplina delle certificazioni mediche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza. La commissione in questione ha condiviso l'affermazione secondo cui la prestazione di cui trattasi non può essere ricondotta, sotto il profilo logico-sistematico, alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, dal momento che non è rivolta, neanche indirettamente, alla tutela della salute dei singoli soggetti o della collettività bensì risponde all'interesse del datore di lavoro pubblico di controllare che effettivamente sussistano le condizioni che giustificano l'assenza dal servizio dei lavoratori.

le certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva sono escluse dai LEA «fatte salve» le prestazioni espressamente indicate nell'ambito dell'attività medico-legale e, tra queste, le «visite di controllo sui lavoratori assenti dal servizio per motivi di salute (visite fiscali) richieste da pubbliche amministrazioni». La modifica avrebbe evitato interpretazioni equivoche e ridotto il contenzioso in atto tra ASL ed amministrazioni pubbliche ma, con ogni evidenza, confermando l'inclusione nei LEA delle visite fiscali, non avrebbe dato seguito all'invito della commissione nazionale LEA di riconoscere la natura peculiare di tale prestazione non rivolta, neanche indirettamente, alla tutela della salute e di individuare modalità diverse per garantirne l'erogazione e per coprirne i costi. Si rammenta, comunque, che sullo schema di provvedimento era stata raggiunta l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il Dipartimento della funzione pubblica, consapevole della rilevanza della questione, ha provveduto a sottoporla ai competenti Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro, salute e politiche sociali, chiedendo se l'orientamento maturato nel passato possa ancora essere seguìto anche a seguito della pronuncia della Cassazione. Per quanto riguarda il Ministero del lavoro, della salute e politiche sociali, posso assicurare che la tematica è seguita con attenzione, alla luce sia della posizione giurisprudenziale della Cassazione sia delle disposizioni introdotte dalla legge n. 133 del 2008. Mi riservo, pertanto, di far conoscere tempestivamente all'onorevole interrogante le determinazioni che saranno assunte congiuntamente al competente Ministro dell'economia e finanze. ringrazio per la risposta che però, mi permetta, è una ricostruzione di un groviglio di competenze

(che, voglio ricordare a tutti, è stato uno dei punti del decreto sbandierato come provvedimento bandiera nella guerra ai fannulloni), non si sono fatte le verifiche necessarie per rendere la norma attuabile. La ricostruzione - la ringrazio per averla fatta così meticolosa - ci dice che si è inserita una norma per decreto sulla quale è stata chiesta la fiducia senza aver verificato chi ne pagava i costi.

senso che alcune scuole che non avevano esaurito i fondi per le supplenze hanno pagato le visite fiscali, altre non le hanno pagate.

penalizzazioni di tipo economico ne risponde in proprio. I dirigenti che, quindi, avevano un minimo di disponibilità in cassa hanno pagato. Mi riferisco alla situazione che conosco, quella della Lombardia, che probabilmente,

una amministrazione pubblica è a carico del Servizio sanitario nazionale, che ha un canale di pagamento del tutto diverso.

una norma chiara e quelle che hanno già pagato devono essere rimborsate. Approfitto di avere la parola per informarla che, peraltro, le scuole, che pure sono enti autonomi come previsto dalla Costituzione, non hanno le risorse per l'ordinaria gestione e il Ministero dell'istruzione ha scritto loro di far pure i bilanci sbagliati, al buio, che pur essendovi il bilancio dello Stato, non è in grado di dire quante risorse darà alle scuole per il loro normale funzionamento. Il risultato sarà che qualsiasi dirigente scolastico non manderà una visita fiscale neanche per sbaglio, e questo è il risultato degli interventi

La causa dell'origine dell'acufene non è chiara. Tuttavia, la ricerca in questo campo sta progredendo e, anche grazie a strumenti innovativi, come le tecniche di *neuroimaging*, che consentono di osservare l'attivazione delle aree del cervello deputate alla elaborazione dei segnali acustici, si stanno acquisendo importanti informazioni sulla relativa eziologia. Dal punto di vista terapeutico, nuove e più efficaci strategie sono in via di sviluppo come, ad esempio, il recente metodo di cura denominato «esposizione a rumore bianco fenestrato», che promette di produrre un sensibile miglioramento della sintomatologia in un lasso di tempo notevolmente inferiore a quello dei trattamenti attualmente disponibili. Con riferimento all'incidenza dell'acufene nella popolazione, in base agli studi condotti negli ultimi dieci anni in Germania, nel Regno Unito e in altre nazioni europee, risulta che mediamente circa il 10-20 per cento della popolazione europea ne ha sofferto almeno una volta nella vita. Studi condotti in Italia su campioni limitati di pazienti hanno dimostrato come anche nel nostro Paese la prevalenza sia analoga e i soggetti che risultano interessati dalla patologia in questione vengono stimati in circa 3 milioni. Tuttavia, da un'analisi della letteratura scientifica, una stima ufficiale della diffusione del problema, effettuata su un ampio numero di individui rappresentativo dell'intera popolazione nazionale, non è al momento disponibile.

modifiche, in quanto nella individuazione delle patologie si è ritenuto che tale condizione non rispondesse a tutti i criteri dettati dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ossia gravità clinica, grado di invalidità e onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo delle prestazioni utili al medico per effettuare un corretto *follow up* della malattia.

del 5 febbraio 1992, recante «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti», che fa riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulle capacità lavorative, prevede tra le malattie invalidanti, al codice 4001, gli acufeni permanenti o subcontinui di forte intensità e insorti da più di tre anni, sia pure con una percentuale di modesta entità. Quanto allo sviluppo della ricerca, questo Ministero, pur riconoscendo l'importanza di tale disturbo, allo stato attuale, tenuto conto delle risorse economiche al momento disponibili, ha inteso negli anni passati privilegiare il finanziamento della ricerca relativa a patologie a

Nel 2009, nell'ambito dei bandi per la ricerca sanitaria, non sono previste tematiche prefissate, pertanto potranno essere presentati e valutati specifici progetti di ricerca sull'acufene.

Signora Presidente, rispondo anche per la senatrice Sbarbati che ha presentato analoga interrogazione. L'acufene, come ha detto il Sottosegretario, è uno dei disturbi più comuni e nello stesso tempo meno conosciuti in Italia. Studi accreditati hanno rilevato che la malattia può insorgere già in età pediatrica, anche se il rischio maggiore naturalmente aumenta con l'età e può raddoppiare dopo i quarant'anni. Naturalmente, come è noto, questo particolare suono fastidioso ha un impatto altamente negativo per quanto riguarda la qualità della vita dei soggetti colpiti, al punto che la persistenza dell'acufene nel tempo interferisce in maniera incisiva nella vita di coloro che ne soffrono. Chi soffre di acufene non riesce a svolgere una vita normale, non soltanto dal punto di vista fisico, ma soprattutto psicologico. Molte persone sono costrette ad un cambio di abitudini che naturalmente va ad incidere sullo stile di vita con l'impossibilità spesso di svolgere attività che richiedono concentrazione, e nei casi più gravi, viene richiesta l'interruzione dell'attività lavorativa o, almeno, il cambio di mansione nell'ambito del lavoro Alcuni dei motivi per cui questa malattia insorge sono i traumi acustici o cranici, a seguito di processi patologici che colpiscono l'orecchio interno, l'assunzione di farmaci ototossici o - dato ancora più grave - nel 60 per cento non è possibile individuare uno specifico fattore scatenante. Se si considera che in Italia i soggetti portatori di acufene siano oltre 3 milioni e che vanno sommati ai 6 milioni di italiani che soffrono di disturbi uditivi di vario tipo di vario tipo ci rendiamo conto di quanto siano alti i costi, che si attestano sui 320 milioni di euro annui per la fascia al di sotto dei 12 anni di 3,3 miliardi di euro annui per le persone al di sopra dei 12 anni per un totale di circa 3,6 miliardi di euro, pari al 5 per cento del fondo sanitario nazionale. Mi riferisco ovviamente a dati che riguardano tutte le persone affette da disturbi dell'udito, a cui non vanno sottratti a questo punto i portatori di acufene.

Rosato rispondeva testualmente che confermava la propria attenzione e sensibilità verso le più idonee iniziative di studio e di ricerca in materia utili ad individuare le terapie più idonee per questa categoria di pazienti.

che vi siano degli studi e delle ricerche su questa patologia, ma in questi anni un granché non è stato fatto. Invece, l'importanza di conoscere questa malattia come grave è la risposta migliore che si può dare oggi ai pazienti che si trovano in queste condizioni. Credo che un intervento da fare subito dovrebbe essere quello volto a finanziare in maniera specifica studi e ricerche scientifiche necessari a dare maggiori risultati ed informazioni in merito a tale patologia. Servono poi azioni in grado di ridurre l'elevato inquinamento acustico ambientale,

importante riconoscere l'acufene come malattia cronica; mi rendo conto che sarebbe forse un passo in avanti eccessivo, ma spero che almeno dal punto di vista della ricerca e delle campagne di informazione e prevenzione sia fatto

sulla relazione della collega che mi ha preceduto, che ha fornito anche un quadro complessivo di quella che abbiamo definito una vera e propria malattia. Tra l'altro, siamo stati anche sollecitati da moltissime associazioni che hanno posto all'attenzione dei senatori della Repubblica questo fenomeno,

sembra un'ipotesi rara ma purtroppo è molto presente, e le posso dire che spesso deforma anche lo stesso apparato uditivo dei ragazzi, per cui diventa quasi impossibile poter vivere normalmente il rapporto

Ringrazio anche l'Associazione italiana Tinnitus-Acufene che sottolinea sempre questo problema, riportando la stima dei pazienti colpiti (oltre

presta una certa attenzione ai disturbi della vista, quelli acustici si considerano sempre «figli di un Dio minore». È quindi importantissimo fare campagne di comunicazione, di sensibilizzazione

Esortiamo il Governo e lei, signor Sottosegretario, a promuovere studi attraverso gli organi di consulenza del Ministero, quale l'Istituto superiore della sanità ed altri, a promuovere ricerca guardando al settore pubblico, ma anche a quello privato che molto spesso può essere di ulteriore volano,

La seduta è tolta